nei primi giorni dello scorso mese di novembre e in conformita a quanto comunicato dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente quanto segue. In seguito alle eccezionali avversita` atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2010, la Regione Basilicata, in data 26 gennaio ha inviato, al dipartimento della protezione civile, un censimento dei Comuni interessati, a disposizione dell’interrogante, con i relativi danni e necessitaeconomiche. Sulla base di quanto comunicato si rappresenta che tali danneggiamenti riguardano, in larga parte, strade comunali. Infatti, sia nella provincia di Potenza che in quella di Matera, sono stati segnalati dissesti della sede stradale che hanno impedito l’accesso ad insediamenti urbani, produttivi e rurali con danni per complessivi 9 milioni di euro. Di questi, circa 1 milione di curo riguardano i danni relativi ai dissesti su strade provinciali e statali, mentre un altro milione e mezzo di euro sono relativi ai danneggiamenti di sponde, argini fluviali e alvei occlusi dai fenomeni franosi delle sponde stesse. In tale contesto sono stati evidenziati solo due eventi particolari: il primo, nel comune di Grassano, in provincia di Matera, che riguarda l’allagamento del centro urbano con un rischio per la pubblica incolumita, e il secondo nel comune di Bernalda, sempre in provincia di Matera, relativo alla rottura degli argini del fiume Bradano. Quest’ultimo evento ha danneggiato le strade comunali di accesso agli insediamenti abitati, agricoli e zootecnici e ha interrotto la linea ferroviaria Taranto-Crotone, interessando 250 persone. Dai dati trasmessi non erisultata la sussistenza di significative situazioni di pericolo incombente sui centri abitati e sulle infrastrutture di primaria importanza, quindi si e ritenuto che tali interventi potessero essere ascritti ad eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225 del 24 febbraio 1992. Ciononostante, data l’elevata estensione del fenomeni che hanno interessato 38 diversi Comuni nelle due Province della Regione e considerata la presenta di eventi come la riattivazione di rischio residuo, si e ritenuto di emanare una norma, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, con la previsione di adeguate risorse economiche, previa l’apertura di contabilitaspeciale. Per quanto attiene alle risorse finanziarie, si fa presente che il 14 dicembre 2010 e stato stipulato l’Accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Basilicata, finalizzato al finanziamento degli interventi urgenti di difesa del suolo, per un totale di 26,935 milioni di euro. Di questi, 20,200 milioni di euro sono stati stanziati dal Ministero dell’ambiente

Si informa, infine, che la Regione Basilicata ha richiesto la dichiarazione di stato di emergenza con le note del 29

nel far fronte agli interventi necessari a restituire funzionalitaalle infrastrutture danneggiate nonche´ ai gravi danni subiti dalle imprese agricole operanti in tale territorio, anche al fine di evitare che le stesse, in mancanza di adeguate misure di sostegno,

che ha messo letteralmente in ginocchio il settore produttivo, in particolare quello agricolo, zootecnico e turistico della Regione Basilicata, soprattutto nella provincia di Matera, con un riverbero nefasto per il reddito delle nostre aziende, e per il quale e stato richiesto il riconoscimento dello stato di calamita. Devo dire che ad oggi, a distanza di circa 9 mesi dall’evento del 2 novembre 2010, l’unico atto

che non estato citato dal Sottosegretario, con il quale e stata dichiarata invece l’esistenza del carattere di eccezionalitadegli eventi calamitosi del 2 novembre 2010 nella provincia di Matera. a seguito di tale decreto, non c’e stata una comunicazione successiva da parte del MIPAF rispetto alle somme disponibili: nessun trasferimento di risorse c’estato in favore della Regione Basilicata. Signor Sottosegretario, credo che non serva dichiarare lo stato di calamita se poi non seguono i fatti. L’unico fatto certo eche, ancora una volta, il nostro comparto agricolo e lasciato solo da

battano un colpo, perche´ fino ad oggi non possiamo non registrare che l’agricoltura non eritenuta un settore strategico, una delle carte vincenti su cui scommettere, un motore trainante della nostra economia. Manca una politica agricola nazionale, manca un piano di rilancio, manca una prospettiva. Signor Sottosegretario, credo che le scelte vadano fatte soprattutto nei momenti difficili, perche´ e in quelli che bisogna individuare le priorita. Credo che sia arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti, di compiere delle scelte, se e vero, come io ritengo, insieme

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche´ delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria

ne´ una prima ordinanza che consenta il rimborso delle spese sostenute dalla Regione e dalle amministrazioni locali per la prima emergenza, ne´ un’ordinanza che, come nel recente caso del Veneto, preveda norme e risorse adeguate per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, per la messa in sicurezza del territorio, nonche´ per il ristoro dei gravi danni subiti dalle imprese agricole, zootecniche e turistiche e, in particolare, per il rilancio del sistema Siamo di fronte ad un grave ritardo dovuto esclusivamente alle particolari nuove, penalizzanti e inique norme emanate con il decreto milleproroghe, che in materia di finanziamenti pubblici, in caso di calamita` naturali, prevede stenografico 21 luglio 2011 E[]di tutta evidenza lo stato di prostrazione del settore imprenditoriale, gia fortemente provato dalla crisi economica; edi tutta evidenza la penalizzazione della nostra Regione rispetto a situazioni, come quella del Veneto, quasi contestuali all’emanazione del decreto-legge n. 225 del 2010; e di tutta evidenza la situazione di necessitadelle amministrazioni pubbliche locali in presenza di un tessuto sociale e produttivo debole, pertanto non suscettibile di ulteriori aggravi di tassazione. ]inaccettabile da parte del nostro territorio il fatto che i costi, non solo della fase emergenziale, ma, a maggior ragione, anche delle opere di ripristino e di ristoro degli ingenti danni, ricadano sulla popolazione lucana, peraltro priva

di competenza statale relativo alla predisposizione e all’attuazione delle ordinanze, ormai non piuprocrastinabile, atteso che comincia a manifestarsi un clima sociale negativo intollerabile, pervaso da un malcontento crescente, prevedendo altresı una deroga alla previsione del milleproroghe per tale evento calamitoso. Credo si tratti di un atto doveroso verso le imprese agricole, zootecniche e turistiche e verso i cittadini delle zone colpite. Se evero, come proclama sempre l’Esecutivo Berlusconi, che il rilancio del Sud e una sua priorita,